l'ordine del giorno della seduta pomeridiana di oggi è stato integrato con il seguito della discussione della risoluzione della 14ª Commissione permanente sul programma legislativo europeo, nonché con l'esame di due ratifiche di accordi internazionali con la Francia e con la Polonia. Resta confermata, per domani mattina, la discussione delle mozioni sulla politica ambientale. Nella seduta pomeridiana di martedì 20 marzo saranno poste all'ordine del giorno le mozioni sull'accattonaggio minorile, sugli ufficiali di Marina in ferma prefissata e sull'industria conserviera del pomodoro.

(qui siamo un po' nel tema della politica europea del nostro Governo), quando è stata deposta la corona sull'Altare della Patria a Roma, il Presidente della Repubblica Slovacca, accompagnato dal ministro Parisi,

Devo ricostruire brevemente le vicende che si sono succedute, altrimenti appare difficile ragionare in maniera corretta di quel che accade. Voglio fin da adesso dire, signor Presidente, che questo richiamo al Regolamento ha soltanto lo scopo di fare in modo che ci sia agli atti una ricostruzione corretta dell'applicazione del Regolamento, affinché qualche anomala interpretazione non costituisca precedente. Il senso è solo questo. Signor Presidente, lei ha chiuso questa mattina i lavori della nostra Assemblea specificando testualmente: «Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con all'ordine del giorno le comunicazioni del Presidente, integrate con le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo». Le ricordo che l'ordine del giorno che era stato ritualmente pubblicato per le sedute antimeridiana e pomeridiana di oggi prevedeva esclusivamente l'Atto Senato n. 1329, ossia il decreto-legge che abbiamo licenziato questa mattina.

È chiaro che tutto questo non è stato fatto. È evidente che la Conferenza dei Capigruppo non può assolutamente violare l'articolo 56, che è dettato nella logica del regolare svolgimento dei lavori e nell'interesse di tutti i colleghi, i quali dovrebbero sapere,

Ci tengo che questa precisazione rimanga agli atti affinché ciò non possa costituire precedente, magari in tempi non di pace come questi, quando vi è una Assemblea che vuole continuare su questo ordine del giorno (e non sarò io ad impedirlo). È un atteggiamento assunto in palese violazione dell'articolo 56, comma 1, del nostro Regolamento, che non è un orpello trascurabile, ma rientra in una logica di sana gestione della dinamica dell'Assemblea che deve essere comunque rispettata.

informata di questo incidente diplomatico (se così lo possiamo definire) ed è intervenuta la mattina successiva organizzando un incontro, che non era calendarizzato, tra il presidente del Consiglio Prodi ed il Presidente della Repubblica Ho notizia della soddisfazione da parte del Presidente della Repubblica Slovacca rispetto a questo tempestivo incontro organizzato dalla Presidenza del Consiglio, che ha in qualche modo risolto positivamente una situazione che conteneva elementi di scabrosità.

sul programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2007 e sul programma di 18 mesi delle Presidenze tedesca, portoghese e slovena***

da un certo punto di vista, strumentale anche rispetto a chi crede. Nello stesso tempo, penso che la questione sia stata già risolta in Europa, perché è chiaro che in Europa dobbiamo mettere insieme

puntano invece non tanto a un'Europa ibrida ma ad un'Europa plurale, diversa e molteplice, come ha detto anche la Merkel, in maniera molto forte; e quando ella ha affermato che l'Europa dev'essere molteplice, diversa e plurale ha detto che la tolleranza è il vero valore su cui fondarsi. Queste sono le motivazioni del mio

Signor Presidente, a nome del Governo esprimo ovviamente parere favorevole alla risoluzione elaborata dalla 14a Commissione, ringraziando anche il relatore, il Presidente e i componenti della Commissione per il lavoro approfondito che è stato fatto.

e che è riferita soprattutto all'attivo contributo dell'Italia alla stesura della Dichiarazione di Berlino del 25 marzo e anche all'idea di sviluppare un'adeguata campagna di sensibilizzazione, indispensabile per rilanciare in positivo i valori dell'integrazione europea nel nostro Paese.

di valorizzare questo ulteriore cammino di rilancio della prospettiva europea. È un'impostazione che ci vede assolutamente favorevoli e che sta impegnando il Governo anche in questi mesi, in questo - devo dire - anche in continuità con le azioni svolte dal precedente Governo. Vorrei ricordare a tal proposito,

legislatura, peraltro in coincidenza con la Presidenza di turno dell'Italia dell'Unione Europea, ha trovato numerose occasioni di discussione in Senato. Anche alcuni dei temi che sono oggetto specificamente degli ordini del giorno ulteriori G2, G3, G4 e G5 sono stati affrontati in quella sede, nonché in sede di Convenzione europea. Fino a poco fa era presente il presidente Dini, che è stato uno dei protagonisti di quella discussione. Alla fine abbiamo convenuto, come Italia, con una larghissima maggioranza parlamentare,

ma anche consapevoli del fatto che nell'insieme alcuni elementi che noi avevamo evidenziato nel corso del dibattito, inclusi quelli sui quali si è soffermato poco fa il relatore senatore Mele, avevano trovato un adeguato accoglimento nel progetto di Costituzione europea.

la bozza di risoluzione che dovrà essere sottoposta all'approvazione del *Summit* di Berlino, emergano qua e là voci dissonanti o tentativi di veto rispetto all'ulteriore cammino di questo progetto. È un lavoro È un lavoro diplomatico molto delicato, che il Governo italiano si è impegnato ad assecondare in tutte le forme, sia per tener fede alla sua tradizione di Paese europeista e tra i fondatori dell'Europa Unita, sia per salvaguardare, in coerenza con i suoi atti parlamentari precedenti e con il voto degli elettori italiani, il più possibile la prospettiva della Costituzione europea. Al Governo sembrerebbe molto inopportuno in una sede come questa inserire, invece, una qualche specificazione, un qualche condizionamento rispetto all'ulteriore cammino, che indebolirebbero l'azione del Governo italiano, in ciò interprete della generalità delle volontà del nostro Parlamento e del nostro popolo, e che probabilmente costituirebbero un ostacolo per la stessa iniziativa del cancelliere tedesco.

dei documenti che noi condividiamo (alcuni li possiamo anche condividere nel loro insieme), il nostro è un invito al ritiro con una riserva che possiamo mantenere. Pertanto, se e quando dopo la Dichiarazione di Berlino ripartirà il processo

l'azione del Cancelliere tedesco e del Governo, di pieno supporto alla stessa, sarebbe lesiva degli interessi del nostro Paese, e soprattutto correrebbe il rischio di vanificare lo sforzo che si sta compiendo. Questa è la ragione per la quale il Governo

ex componenti della Convenzione - cito il senatore Follini, il senatore Dini, il ministro dell'interno Amato - che hanno lavorato attivamente a questo progetto; ora mi parrebbe strano

Signor Presidente, colleghi senatori, l'Aula è oggi chiamata ad esprimere il proprio voto su una risoluzione della 14a Commissione predisposta a seguito di un dibattito approfondito concernente l'azione europea espressa nei due documenti programmatici della Commissione europea. La Commissione ha illustrato un *focus* rispetto alle sfide comuni con le quali l'Europa oggi si confronta e dovrà continuare a confrontarsi con sempre maggiore impegno e coesione: la sicurezza, la globalizzazione, il mutamento climatico, il problema energetico, la politica sociale e tanti altri temi ancora. Per ottenere risultati concreti e, soprattutto, condivisi rispetto alle suddette problematiche l'Unione Europea ha però un altro indispensabile traguardo da raggiungere: il suo completamento politico ed istituzionale. L'*iter* delle ratifiche nazionali per l'esecuzione del Trattato che istituisce la Costituzione Europea, approvato a Roma il 29 ottobre 2004, ha già ottenuto l'approvazione dei due terzi degli Stati e della maggioranza dei cittadini dell'Unione. Gli Stati che non hanno ancora ratificato il Trattato sono impegnati fin dal 29 ottobre 2004 a provvedervi nelle forme stabilite dalle procedure nazionali. E' sempre più evidente l'urgenza di riattivare il processo costituente superando gli ostacoli frapposti dall'esito negativo dei *referendum* in Francia e Olanda, uscendo definitivamente dalla fase di riflessione ormai troppo lungamente protratta. Essenziale a tal fine è proprio la Conferenza dei Capi di Stato e di Governo che si riunirà a Berlino il prossimo 25 marzo nel cinquantenario dei Trattati di Roma, e la Dichiarazione che si attende in quella circostanza. Il Governo italiano in quell'occasione sarà chiamato a fornire ancora una volta il suo prezioso contributo nel processo costituzionale europeo, ed è proprio in tal senso che oggi il Senato vuol impegnare l'Esecutivo, ponendo l'attenzione in special modo su un aspetto fondamentale per la realizzazione dei processi di integrazione. Occorre adoperarsi concretamente per lo sviluppo di una sensibilità europea soprattutto nelle nuove generazioni, sensibilità europea intesa quale sinonimo di condivisione delle ragioni dell'Unione, condivisione dei valori dell'Unione, valori comuni e realmente sentiti come propri dal cittadino europeo, in assenza dei quali ogni tentativo di riforma risulterà vano.

desidero condividere anche gli accenti positivi e quasi entusiastici con i quali la ministra Bonino ieri sera ha commentato il tenore, il tono, il livello del dibattito che si è sviluppato su questo tema; un tono che sicuramente è andato al di là della ritualità e mi piace immaginare che questo rinnovato entusiasmo verso temi che solitamente sembravano consegnati all'impegno degli addetti ai lavori sia motivato dalla vicina scadenza del 25 marzo e quindi dell'impegno che attende ritualmente tutti noi a Berlino. Se potessi indirizzare una raccomandazione a coloro che avranno la responsabilità di scrivere questa dichiarazione sull'Europa a Berlino, consiglierei loro di celebrare certamente i meriti di chi fondò l'Europa e di chi la costruì, quindi del passato, di celebrare indubbiamente la nostra storia, ma di avere la capacità, subito dopo, di alzare l'orizzonte e guardare verso il futuro. Da Berlino ci aspettiamo, infatti, soprattutto una spinta in prospettiva il futuro direi che è ben disegnato in questo momento di riaccesa attenzione su temi comunitari proprio dalle conclusioni che il dibattito ha portato e dalla sintesi del documento. È vero, forse ha ragione il senatore Manzella, esso è un po' troppo stringato, inevitabilmente sintetico, ma credo sufficientemente indicativo dei sentimenti, se non di proposte concrete che possiamo passare. Ebbene, direi che anche l'evento nuovo ed inedito che tre Presidenze, quella tedesca, quella portoghese e quella slovena, si siano messe d'accordo per concordare un programma comune di 18 mesi è un buon segno, c'è quindi aria nuova in Europa ed è questa aria nuova che si dovrebbe seguire a Berlino. E soprattutto le priorità sono indicative di una evoluzione che fortunatamente c'è: per esempio, il completamento inevitabile, necessario della Strategia di Lisbona nelle dimensioni dello sviluppo economico, delle riforme sociali, dell'attenzione per l'ambiente e poi l'ampliamento ed una maggiore tutela dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, soprattutto con l'impegno vero e concreto dei Paesi membri verso la lotta al terrorismo, la lotta ai trafficanti di droga e di esseri umani. E poi questo tanto agognato ruolo esterno dell'Unione, una vera e propria - auguriamoci - politica estera che dovrebbe realizzarsi sempre verso la sicurezza e lo sviluppo, ma anche verso le relazioni economiche, il tutto proiettato fino all'ultima delle nuove frontiere che il coraggioso allargamento del 2004 aveva portato, nuove frontiere soprattutto verso Est. Ancora, le iniziative annunciate nel programma del Consiglio verso la promozione dell'integrazione europea, soprattutto nelle scuole, fino a un'interessante annotazione sul cambiamento demografico demografico che è in atto in Europa in due direzioni, che non sono opposte, ma camminano parallelamente: una specie di staffetta generazionale tra gli anziani

la valorizzazione economica e la riattualizzazione della persona anziana anche per il valore economico che ancora può rappresentare.

coerenza anche con l'ultima evoluzione che si è avuta verso Est. Su quasi 450 milioni di abitanti di cui oggi dispone l'Unione Europea, più del 20 per cento sono giovani e hanno meno di 30 anni. È a questi che che dobbiamo consegnare una staffetta, non solo ideale, con il documento di Berlino. Il potenziale c'è. C'è una novità in più: molti di questi giovani appartengono ai Paesi dell'Est e sono alle prese con un'esperienza indubbiamente nuova ed entusiasmante per loro, quella di una democrazia riconquistata in maniera totale. Sono Paesi in cui ancora si vedono la disoccupazione, proprio nella fascia giovanile, il divario del prodotto interno lordo, la scarsa meccanizzazione dei settori produttivi e il limitato potere di acquisto sono dislivelli che molti di questi *partner* sono ancora impegnati a colmare. Su

l'aspetto non secondario di un disegno complessivo, nel quale appare chiaro come solo in un'Europa delle eguaglianze potranno realizzarsi condizioni di reale democrazia e potrà trovare alimento ideale la diffusione della dottrina cristiano-sociale, tema che interessa la mia parte politica e che nel Partito popolare europeo - di riferimento sempre per la mia parte politica costituisce la frontiera ideale irrinunciabile per qualsiasi sviluppo. La cornice del suddetto disegno sarà il recepimento della Carta costituzionale europea nel maggior numero possibile di Paesi membri: una Costituzione forse ancora debole - questo è vero - nel ribadire le comuni radici religiose, i diritti fondamentali del cittadino, conclamati nella Carta di Nizza, e debole sul piano della difesa della famiglia, del diritto al lavoro, alla casa, a un'occupazione, all'istruzione

europea. Certamente si poteva pretendere una Carta più coraggiosa, ma in Europa si è sempre proceduto per piccoli passi e in quel momento storico e in quelle condizioni è il massimo che si potesse immaginare. È un segnale promettente anche per chi crede nell'etica come valore base dell'impegno politico del cittadino. Diceva Alexis de Tocqueville: «L'uomo non può godere della libertà politica se non a prezzo di molti sacrifici e la ottiene sempre e solo con grandi sforzi». De Tocqueville ci aveva consegnato anche un'altra massima, molto attuale per i Paesi di recente libertà.

«l'uomo deve imparare a comprendere quanto sia stretto il legame del suo vantaggio personale con quello della collettività» Ecco, quindi, i valori morali che si innestano sui valori materiali e economici che ho indicato prima. In questo campo è utile non dimenticare

sono le pietre miliari della nuova Europa». Diceva, ancora: «La vita senza responsabilità politica è certamente più facile, soprattutto nel disordine attuale. Ma nessuno ha il diritto di sottrarsi alle sue responsabilità.

E allora, Presidente, non possiamo mentire a noi stessi: la strada verso l'integrazione europea indubbiamente è ancora molto lunga, ma se i Paesi membri non recepiranno la Carta costituzionale, questa strada sarà inesorabilmente sempre in salita.

alla risoluzione, volevo ringraziare i senatori Mele e Manzella per l'ottimo lavoro, nonché il Governo per l'entusiasmo europeista. Signor Presidente, è noto che il quarto movimento «Allegro con brio» della nona sinfonia di Beethoven è l'inno ufficiale dell'Unione Europea.

Nietzsche - nel senso che oggi lo *show* e la vita sono fatti tutti con le contaminazioni e probabilmente anche la biopolitica odierna è figlia di quest'idea wagneriana dello spettacolo totale in cui le contaminazioni si ripetono.

A parer mio queste parole dovrebbero essere, e sono, pace, democrazia, ambiente, lavoro e diritti. Sulla pace non mi soffermo, perché davvero credo che già il processo costitutivo dell'Unione Europea sia di per sé uno degli atti fondativi di pace di questo pianeta più interessante e più intelligente mai verificatosi nella storia. e di collaborazione in un territorio e in una determinazione geografica che è sempre stata il nucleo di tutte le più grandi tragedie di questo pianeta (penso ad Auschwitz, alla Prima e alla Seconda guerra mondiale,

davvero nella storia dei popoli. E sottolineo che Prodi, probabilmente, sarà ricordato nella storia proprio per la forzatura su questo allargamento,

Sulla pace, aggiungo solo che mi spiace non si sia riusciti ad includere, all'interno della Carta dei diritti fondamentali dell'Europa, l'articolo 11 della nostra Costituzione; però già il processo europeo in sé è davvero un atto di pace.

è indubbio che vi sia un *deficit* di democrazia, di partecipazione e di chiarezza sulle responsabilità e sulla rappresentanza. Penso si debba fare di tutto - com'è nella norma democratica e nella civiltà giuridica che dal 1600 in avanti ha sostanziato il nucleo della rappresentanza

In questo processo, la questione del Trattato costituzionale - su cui, onestamente, abbiamo avuto molte critiche e perplessità,

connessione di Stati e poteri forti, mentre troppo poco come espressione di contaminazioni, non solo di Stati, ma di regioni, bioregioni ed etnie diverse, che scommettono forte sul fatto che, in questo pianeta, l'unica possibilità per andare avanti è appunto convivere e trovare le forme per le decisioni e la sussidiarietà comuni. La terza questione che intendo

sui propri rifiuti e inceneritori, in un'espansione totale, per cui una megalopoli diventa solo rifiuti e nient'altro - è un altro dato che può porre l'Europa

agli agglomerati degli altri Stati, penso agli Stati Uniti. È indubbio però che in Europa vi è un'erosione dei diritti del lavoro, un'erosione del lavoro in sé - sono riflessioni sulla globalizzazione e sulla produzione indubbio che sia necessario, da una parte, avviare una grande stagione con sindacati europei all'altezza delle sfide e dall'altra, recuperare una capacità europea di interagire con la globalizzazione

sul pianeta in tema di difesa dei diritti. Concordo pienamente sulla questione dei diritti in politica estera

la risoluzione proposta dalla 14a Commissione permanente per i rapporti con l'Unione Europea, volutamente generica, sconta - è necessario dirlo - pericolose dimenticanze. Sono ineccepibili gli elementi che si vogliono sostenere: democrazia, coesione sociale, progresso economico. Si continua però a parlare in questo modo di un'Europa al minimo denominatore. Almeno qui, in quest'Aula, signor Presidente, dovremmo avere il coraggio di scrivere, nero su bianco, in un documento ufficiale, che prima dell'economia vengono l'identità e la cultura, che vogliamo un'Europa più attenta alle specificità, alle tradizioni e al fondamento cristiano. Ripeto, la Lega Nord condivide le premesse della risoluzione, ma l'impegno non è in linea con ciò che davvero riteniamo importante, prima di tutto perché per noi la Costituzione europea non è un obiettivo da raggiungere a tutti costi. La Costituzione può essere uno strumento ma non un obiettivo e una Costituzione arida, burocratica ed elefantiaca come quella sul tavolo non può assolutamente incontrare il nostro consenso, né, vista la risoluzione, pare ci siano opportunità di miglioramento. D'accordo sulla democrazia e sul progresso economico, ma una Costituzione deve avere un respiro ben più ampio, deve parlare di radici, le radici cristiane d'Europa, di popoli, di identità, di rispetto e di valorizzazione di tali identità. È stato scritto, ad esempio, che vogliamo rispetto ambientale, ma l'ambiente non è un'entità astratta, globale, è amore e tutela del territorio, paesaggio, ritmi di vita, strutture sociali e tradizionali che vivono in simbiosi con l'ambiente da cui derivano. Nessun elemento è scisso dagli altri e la visione europea deve tener conto insieme di tutte queste dimensioni per non sviluppare ricette e soluzioni a compartimenti stagni che creano problemi a catena. C'è un altro tema che ci sta a cuore e vorremmo che fosse maggiormente approfondito; tema al quale la risoluzione non fa cenno, se non forse in via incidentale quando si parla di sicurezza. Il programma di lavoro della Commissione sembra esprimere la volontà ferma di arrivare ad una gestione comunitaria ed europea del fenomeno dell'immigrazione. Il testo parla di vere e proprie, e quindi vincolanti, iniziative legislative. Ma questa idea prospetta buone possibilità e pericolosi rischi. Siamo Paesi di frontiera e di sbarco. Abbiamo bisogno di aiuto, anche finanziario, nella gestione dell'immigrazione ed è interesse dell'Europa che tale gestione sia ordinata, ordinata, stante che molta immigrazione che passa dall'Italia è diretta al Nord-Europa. Ma la materia è difficilissima e come Lega Nord saremo attentissimi agli sviluppi che il diritto di Bruxelles seguirà nel prossimo futuro. sappiamo che la possibilità di incidere da parte parlamentare sulla normativa dell'Unione Europea è ancora limitata e passa in larga parte attraverso l'indirizzo del Governo. Il problema è che, soprattutto in materia di immigrazione, di questo Governo non ci possiamo proprio fidare. Non manca provvedimento che passi da quest'Aula, nel quale non si cerchi di infilare qualche porcata che vanifica la legge in vigore in materia di immigrazione, senza riguardo per il Regolamento del Senato, per l'auspicabile omogeneità in materia di un provvedimento e, soprattutto, senza il coraggio e la trasparenza di proporre una legge di riforma organica ed autonoma; chiaramente perché essa sarebbe un risultato impossibile in una coalizione in cui non si fa niente per non rischiare di litigare. Aspettiamo dunque la normativa comunitaria, sperando che faccia meno danni di una qualsiasi legge di questo Governo sull'immigrazione, come le ipotesi formulate nelle ultime ore. Sperando poi che non si colga l'occasione, al momento di recepirla nella normativa interna, per aggiungere ritocchi qua e là che vanifichino ogni controllo e devastino il Paese. Signor Presidente, per questi motivi l'impegno di questa risoluzione ci sembra vacuo, se non addirittura fuorviante, e la Lega Nord esprimerà voto contrario.

alla vigilia dell'incontro di Berlino che deve rilanciare l'idea europea. So che in Germania è in corso, da parte della Presidenza tedesca, un grande sforzo per andare nuovamente alle radici e alla visione fondamentale dell'Europa, per tentare di costruire un nuovo europeismo. Sono stato qualche mese fa al Kuratorium dell'Adenauer Stiftung presso Jagsthausen e si è messo a punto un grande programma per ridire le ragioni dell'Europa. L'Europa non è cosa delle banche e dei banchieri, non è cosa delle burocrazie di Bruxelles; l'Europa è cosa dei popoli, è l'ideale fondamentale europeo, l'ideale della pace: mai più la guerra in Europa. È da qui che è nata l'idea dell'Europa. E poi la geniale intuizione successiva: il mercato al servizio della pace. Costruire un mercato comune europeo come condizione perché gli europei si facessero concorrenza tra di loro attraverso il commercio, le arti, l'industria, la scienza, non attraverso gli armamenti e la guerra. È molto pericoloso dare questo per acquisito. Dobbiamo ricordare che se venissero meno gli strumenti che abbiamo messo in piedi potremmo tornare in una situazione in cui la guerra tornerebbe ad essere possibile in Europa. Non è vero quello che dice un'ideologia buonista dominante, che la guerra è una cosa strana, straordinaria e la pace è la normalità della vita umana. È vero il contrario: la storia porta naturalmente verso la guerra; la pace è il risultato di sforzi intelligenti, di politiche indovinate, di una continua tensione morale. Dobbiamo rilanciare questa idea Noto con piacere che nella risoluzione che ci viene proposta è accentuato il tema che anche l'Italia dovrebbe avere una grande campagna per dire le ragioni dell'Europa. Questo non implica un europeismo di maniera che dice che tutto va bene. La polemica contro l'eccesso di burocrazia dell'Unione Europea, la polemica contro un Parlamento che a volte parla di tante cose che non sono di sua competenza e non fa bene le cose che invece sono di sua competenza, la sottolineatura del principio di sussidiarietà, secondo cui l'Unione non deve fare quello che fanno meglio gli Stati, o addirittura le Regioni: questo non nasce da antieuropeismo, anzi, è la condizione del nuovo europeismo. Per avere un rilancio dell'idea europea dobbiamo avere la capacità anche di criticare con coraggio alcuni aspetti delle Istituzioni europee, così come si sono venute configurando. Non è possibile rilanciare l'idea dell'Europa senza parlare di cultura, di una famiglia di Nazioni, di radici culturali, le radici cristiane (o, meglio, ebraico-cristiane), le radici greco-latine, da cui deriva questa famiglia di popoli, altrimenti non si capisce perché l'Europa è quello che è. Dobbiamo avere il coraggio di tornare a parlare di radici. Per questo mi stupisce che il Governo rifiuti il suo assenso ad un ordine del giorno che parla di radici cristiane Credo che se la Germania ha oggi il coraggio di rimettere sul tappeto questo tema l'Italia non può rimanere indietro. *(Applausi dai Gruppi UDC e FI).* Non capisco le ragioni per cui il Governo italiano non si impegna a sostenere l'iniziativa tedesca per rimettere al centro il tema delle radici cristiane dell'Europa, come non capisco le ragioni per le quali in questo momento, invece di lanciare anche in Italia una grande campagna culturale, si parla di abbattere quei pochi strumenti che abbiamo - il Cide, per esempio -, che avrebbero la funzione istituzionale di fare informazione per l'Europa, di spiegare l'ideale europeo, di rilanciare l'ideale europeo. Se c'è un momento di stasi in cui, da parte del Governo, non c'è alcuna iniziativa di promozione dell'idea dell'Europa è esattamente questo. Si capisce il perché: non avendo una prospettiva culturale condivisa lungo la quale parlare di Europa, meglio non parlarne. Nella gente si consolida così l'idea che l'Europa sia un'altra cosa. Credo che nel rilancio sia necessario avere una visione forte e degli obiettivi chiaramente delimitati. Dobbiamo inoltre tornare davanti all'elettorato francese e olandese e ottenere il loro consenso. Signor Sottosegretario, il *referendum* va fatto in Francia e in Olanda! Un *referendum* in tutta Europa non serve a nulla. Le pare mai che la Francia accetterebbe di chinare il capo davanti ad una maggioranza che fosse però minoranza in Francia? Sarebbe la ricetta sicura per mandare in rovina lo sforzo di costruzione europea. Siamone consapevoli. Quello che serve, invece, è la capacità di tornare davanti all'elettorato francese. Bisogna avere una prospettiva culturale chiara, bisogna dire una parola chiara sui confini dell'Europa. L'idea dell'ingresso della Turchia nell'Unione Europea è una delle ragioni fondamentali per cui abbiamo perso il *referendum* in Francia e in Olanda. L'Europa deve avere dei confini. Tutto ciò che ha un'identità ha anche dei confini. Non voglio affrontare in questa sede il tema, complesso, dell'ingresso della Turchia nell'Unione Europea. Devo dire però due cose. La prima è che, quando si comincia dicendo che la religione non è un problema, si comincia con il piede sbagliato. La religione è un problema, perché la cultura è la base dell'Unione Europea. Poi, il problema può forse essere superato, ma non parlarne e far finta che non ci sia è il modo sicuro perché il problema non venga affrontato

illuso e ingannato un popolo orgoglioso, di grande cultura, coraggioso e che merita maggiore rispetto: il popolo turco. A parte questo, però, l'Europa in questo momento chiede un momento di pausa sull'allargamento, non solo riguardo alla Turchia, ma in generale. Abbiamo fatto molto in poco tempo e oggi gli elettorati di tutti i Paesi europei guardano con grande diffidenza a qualunque allargamento. Dobbiamo insistere sui Balcani perché ne va della nostra pace e della nostra sicurezza. Oltre quello, diamoci una moratoria: per un po' di tempo abbiamo il coraggio di dire che di allargamenti ulteriori è meglio non parlare. Io credo che dobbiamo anche domandarci perché l'elettorato francese e olandese ha votato no. Un motivo è stato la mancanza di confini; un motivo è stato una Costituzione farraginosa, troppo lunga, di 437 articoli. Non è possibile. La terza parte va lasciata fuori. La terza parte non serve. Nessuna Costituzione regola nel dettaglio le politiche che fa un Paese. Le politiche andranno regolate secondo quel che sarà il libero svolgimento dei rapporti di forza politici nei Paesi tra i Parlamenti.

negli ultimi tre articoli ha una clausola di autoffondamento, cioè non si applica. Ricordo che li impose la Gran Bretagna. Gli ultimi tre articoli dicono con chiarezza che, nei rapporti comuni tra i cittadini, quella Carta non si applica. Generano però molti equivoci, poiché c'è gente che in Francia ha votato contro la Costituzione perché convinta che la Carta imponesse alla Francia il matrimonio *gay*; e c'è gente che ha votato contro la Costituzione perché convinta che la Carta imponesse di non fare il matrimonio *gay*. In realtà non è vera né l'una né l'altra cosa, perché le politiche familiari sono di esclusiva competenza degli Stati nazionali. E anche questo va detto, perché toglie un altro elemento di difficoltà negli elettorati verso l'Unione Europea. Signor Sottosegretario, non capisco perché il Governo rifiuti di approvare un ordine del giorno che dice queste elementari verità: le politiche familiari e la definizione di cosa sia famiglia appartengono esclusivamente agli Stati membri. Non è una proposizione rivoluzionaria. Voglio rassicurarla, c'è nei Trattati; non solo, c'è nelle dichiarazioni della Presidenza tedesca; solo, c'è nelle dichiarazioni della Presidenza tedesca; non solo, c'è nell'introduzione alla risoluzione che voi ci proponete di votare. E se lo scrivete nell'introduzione, che paura avete di prendere un impegno perché questa verità elementare venga accettata e riconosciuta?

le politiche della famiglia e la definizione di cosa sia la famiglia sono di competenza degli Stati nazionali; vogliamo ripartire dalle radici cristiane dell'Europa.

di poter far intervenire in dichiarazione di voto senatori che invece intendono intervenire sugli ordini del giorno, la Presidenza ha deciso di procedere con le dichiarazioni di voto e il voto sulla risoluzione e poi

GAGLIARDI *(RC-SE)*. Signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, Rifondazione Comunista voterà a favore di questa risoluzione molto generale. Sarebbe stato forse più apprezzabile un documento che impegnasse il nostro Governo in modo più concreto sul tema. In ogni caso, apprezziamo molto le intenzioni positive e simbolicamente rilevanti di questo documento e lo votiamo con convinzione. Dunque, l'occasione che ci è proposta da questo voto resta quella di ragionare sull'Europa, un tema che non è così presente nella nostra discussione, nella nostra ricerca e nel nostro confronto politico come meriterebbe. Vorrei fare solo una premessa di carattere politico complessivo. Credo che l'Europa di cui periodicamente parliamo abbia di fronte a sé un'alternativa molto precisa, molto netta: precisa, molto netta: o sarà un Continente e un grande nuovo Stato, una grande nuova Confederazione di popoli, ricca di autonoma soggettività politica, o non sarà. Credo che questo sia un punto che meriterebbe anche da parte mia una argomentazione più forte, ma credo che la ragione vera per la quale noi scontiamo molti anni di di difficoltà europea ad intervenire ed a giocare un ruolo significativo nei grandi conflitti che si sono aperti - spesso niente meno che nel cuore dell'Europa - nasca dall'assenza di dall'assenza di autonomia politica. Non solo, quindi, siamo di fronte ad una questione di identità da definire con maggiore chiarezza, ma siamo di fronte prima di tutto ad un problema di autonoma soggettività politica e civile. L'Europa è difficile ad essere definita in termini schematici. E' un luogo nel quale si sono inseguite e succedute mille culture e mille momenti di fondazione culturale. Una cosa però è sicura: esiste ormai - ed è questo che vorrei proporre alla vostra attenzione - una cosa che possiamo definire un modello di civiltà europea, un insieme di culture, una disposizione all'incontro tra i popoli, una capacità di essere luogo dell'accoglienza, di di essere anche una sedimentazione seria e profonda di diritti e tutele sociali, che configurano una civiltà europea diversa, identificabile con nettezza. i pensatori neoconservatori americani dicono, come Robert Cogan, che gli Stati Uniti hanno Marte nel loro segno astrologico; l'Europa ha Venere come suo riferimento simbolico. Gli Stati Uniti sono un popolo guerriero; l'Europa è affannata ad inseguire modelli di tutela sociale ed avanzamenti di tipo progressivo per per le sue popolazioni e quindi, in sostanza, rifiuta il suo compito di forza. È un Continente imbelle, dice Cogan. Credo che questa definizione, un Continente imbelle, cioè non dedito alla guerra, che dopo secoli di lacerazioni fratricide e dopo gli orrori della Seconda guerra mondiale ha scelto, forse, di essere imbelle (sceglierei ancora più a fondo questa entità: mi piacerebbe una Europa disarmata; uso questo termine ormai desueto, caduto dal nostro lessico: un'Europa disarmata e comunque imbelle), credo sia il primo tratto forte della identità che noi possiamo dare a questa Europa da rilanciare. da rilanciare. La seconda parola d'ordine che vorrei citare è quella dei diritti, per tutte le ragioni schematicamente accennate prima; parlo di diritti sociali, ma anche di diritti civili, di allargamento di libertà. Se pensiamo che una modesta proposta sulle unioni civili, come quella che impegna in questo momento il nostro dibattito in Europa, è realtà consolidata e tranquilla da molti anni, forse il riferimento europeo che facevo al modello europeo ci può essere utile. Terzo elemento portante per me è la conoscenza: Lisbona è un punto di riferimento per tutti ed anche un punto di riferimento del lavoro di indirizzo di tutti i Governi e segnatamente del Governo della Comunità Europea. Ho sottolineato già molte volte anche in Aula - sembra quasi una fissazione personale, ma lo voglio ripetere qui - che la conoscenza nell'era definita dell'economia della conoscenza è considerata, credo, da tutti gli analisti il motore fondamentale non solo per la diffusione e una democrazia di sostanza, non solo per una capacità dei popoli di controllare lo straordinario sviluppo della scienza e della tecnologia, ma la condizione di base per quelli che continuiamo a chiamare sviluppo e crescita. Non esiste forza economica o crescita senza un grande investimento nella conoscenza, che - ripeto - è anche investimento in sostanza democratica. Infine, sottolineo anch'io, come il collega dei Verdi che mi ha preceduto, la centralità delle tematiche ambientali. Quando parliamo di ambiente non parliamo, come forse si intende, di qualcosa di irenico, del rapporto uomo‑natura in termini opzionali o lussuosi; parliamo di modelli di sviluppo, parliamo di fonti di energia, parliamo di come si organizza, e attorno a che cosa, la crescita economica e sociale di un Paese. In un'era caratterizzata dal rifiuto o dalla non applicazione di una proposta modesta come il Protocollo di Kyoto,

sperimentare non una banale tutela dell'ambiente, ma una capacità di sviluppare politiche di difesa della specie umana e di salvaguardia di questo Pianeta rispetto alle generazioni future. Da questo punto di vista, sono apprezzabili le ultime decisioni europee. Credo e spero che ciò non costituisca la premessa per il ritorno all'uso di quell'energia nucleare che i maggiori Paesi hanno rifiutato,

dei *referenda* in Francia e Olanda. Leggiamo in quel voto, signor Presidente, non il rifiuto dell'Europa, non soltanto, certamente, la lontananza che i popoli avvertono di fronte a un'istituzione ancora troppo lontana; abbiamo letto e continuiamo a leggere in quella bocciatura la domanda di un nuovo e diverso europeismo. In questo senso anche noi di Rifondazione Comunista siamo europeisti convinti. Il problema non è più se fare l'Europa, ma quale Europa e come: se sarà davvero l'Europa dei popoli o l'Europa dei mercati. Grazie. onorevoli colleghi, il dibattito di ieri, per chi lo ha seguito, è stato molto ricco di differenze, di valutazioni e di scale di valori riguardo all'Europa, che provavano come, pur avendosi i medesimi obiettivi, tra le varie parti politiche ci siano ragioni e motivazioni diverse. La risoluzione della 14a Commissione, alla ricerca doverosa del maggiore consenso, che addirittura si è tradotto nell'unanimità alla sottoscrizione della risoluzione stessa, tradisce quello che poi è la cultura europea, che per voler giustamente acquisire il massimo del consenso si accorda sul minimo comune denominatore e quindi su una serie di affermazioni condivisibili, ma nelle quali ognuno trova una parte che in fondo non lo soddisfa o quanto meno non lo soddisfa completamente. Credo che proprio in questo ragionamento ci sia una prima valutazione da fare su questa Europa che stiamo costruendo. Vi è, infatti, il dubbio che l'Europa dell'unanimità dei 27 su molti atteggiamenti, l'Europa che deve cercare a tutti i costi il consenso su ogni singolo atto probabilmente tradisce anche una lentezza, un approccio molto difficoltoso alla risoluzione dei problemi e quindi sostanzialmente un rallentamento nel processo europeo. processo europeo. Voteremo ovviamente a favore della risoluzione della 14a Commissione, che è un po' il mandato che diamo al Governo per le celebrazioni che si terranno a Berlino il 25 marzo,

per largo consenso e quindi con grande attenzione, attenti alle differenze, alle sensibilità e sostanzialmente, come dice Angela Merkel, a una ricerca dell'anima dell'Europa. Allora, in aggiunta al voto favorevole alla risoluzione, esprimo qualche commento sul parere contrario del Governo sugli altri ordini del giorno. Francamente, quando sentiamo affermare questo bisogno di anima, di una forte volontà di partecipazione dei cittadini europei alla costruzione dell'Europa,

maggioranza. Secondo noi, l'Europa non nasce né con il Patto di Nizza, né con la Costituzione. Secondo noi l'Europa ha una storia lunghissima, viene dall'eternità, ha costruito la sua cultura, le sue radici, la sua storia, si è così conformata attraverso terribili guerre civili, scontri di religione, nelle differenze profonde delle culture. Oggi, ridurre questa Europa a un patto tra giuristi e avvocati francamente estremamente riduttivo. Accentuo questo aspetto perché non capiamo la difficoltà che hanno questa maggioranza e questo orientamento politico ad accettare il concetto di difendere le radici cristiane dell'Europa. Nessuno, credo, almeno da parte nostra, vuole invocare oggi un'Europa che debba trovare nel magistero della Chiesa il suo punto di riferimento, ma noi affermiamo che l'Europa, in quanto tale, per come si è costruita, ha nella storia e nella cristianità il suo *humus* e la sua unità. Quando discutiamo, ad esempio, del rapporto con la Russia, se la Russia faccia parte o meno dell'Europa, qual è il tema se non quello di riconoscere che la Russia è una grande potenza cristiana, che la religione cristiana-ortodossa è, nella sua

banchi del Governo - che questa è l'Europa della democrazia e dei diritti, è poco. L'Europa non è costruita solo nel nome della democrazia, perché democrazia e diritti sono il risultato della storia dall'Europa. Come si fa a dimenticare che la separazione tra Stato e Chiesa è un processo culturale sviluppato in Europa e nato in accordo tra il Sacro romano impero e la Chiesa cattolica? Senatrice Menapace, credo di poter affermare che uno dei più grandi Stati laici era il Sacro romano impero di Francesco Giuseppe, imperatore d'Austria, a cui va la mia memoria e il mio riconoscimento.

Come fa l'Europa oggi a proporsi nel mondo dimenticando il diritto romano, la storia di Roma, la cristianità di Roma? Allora, perché cercate un'anima? Ma dove la cercate quest'anima? Jacques Delors è l'uomo delle procedure, un grande europeo. Ci insegnò che attraverso i regolamenti, le procedure, l'abitudine a stare insieme si poteva costruire anche questa Europa. Ma l'Europa di Jacques Delors è senz'anima. Non ha, voglio dire, lo spirito, la volontà, la partecipazione dei cittadini. A cosa partecipano?

non possiamo accettare che il Governo respinga gli ordini del giorno in cui vi chiediamo, perlomeno, di impegnarvi insieme ad altri Paesi, soprattutto vista la nuova posizione che ha assunto la Germania, per ribadire questo concetto. Mi domando ancora di più se senza radici cristiane è l'Europa della laica Francia, nella quale è negato per legge fare manifestazione della propria fede, sia nel portare la croce latina sia nel portare il velo. Ebbene, noi vi diciamo no, no, non è questa l'Europa che vogliamo costruire, un'Europa cioè che non abbia l'orgoglio dei propri valori, della propria fede e della propria storia. Signor Presidente, mi avvio a concludere. Noi voteremo a favore della risoluzione della 14ª Commissione,

primo firmatario il senatore Zanone, voteremo a favore dicendo con grande sincerità che forse, più che di *referendum* e di atti che alla fine diventano solo atti formali e che poco aggiungono alla vicenda dell'Europa,

Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole di Forza Italia alla risoluzione che è oggi all'esame del Senato siamo consapevoli e preoccupati della lunga *impasse* nella quale versa da qualche anno il processo di adesione dei 25 Stati membri al Trattato di Costituzione europea firmato a Roma il 29 ottobre 2004, siglato per l'Italia dal presidente della Repubblica Ciampi e dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Ma secondo il Trattato di costituzione UE, ancora vigente, il voto contrario di anche uno solo tra i Paesi membri ha il potere di interrompere l'intero processo decisionale. Tale disposizione non permette quindi, allo stato attuale, a seguito dei fallimentari *referendum* svoltisi in Francia e in Olanda, di uscire dall'*impasse* nella quale è precipitata l'Europa nonostante le prolungate pause di riflessione che scadranno però nel giugno prossimo. Per chi non lo ricordasse, dei 25 Paesi il Trattato è stato ratificato da 18 (tra cui l'Italia), è stato bocciato da 2 (Francia e Olanda) e hanno interrotto la procedura di ratifica in 7. La speranza di poter sbloccare questa difficile situazione di stallo è riposta soprattutto nel semestre di presidenza tedesco, cominciato nel gennaio di quest'anno e che, nel programma titolato «Realizzare l'Europa insieme» ha riportato la centralità del rilancio del Trattato costituzionale. Al primo posto dell'agenda del cancelliere tedesco Angela Merkel c'è proprio la ricerca di una soluzione condivisa che consenta di uscire dall'*impasse*. Dalla Dichiarazione di Berlino del prossimo 25 marzo, celebrativa del cinquantesimo anniversario dei Trattati di Roma, al Consiglio europeo del giugno 2007, la Presidenza tedesca fisserà i paletti di questo rinnovato percorso, con l'approvazione di una *road map* per il varo di tale necessaria riforma istituzionale entro le elezioni europee del 2009. Non sarà facile per la Merkel, come per nessuno Stato membro di questa Europa, che è oramai formata da 27 Paesi con esigenze ed aspettative tanto diverse, produrre decisioni in un regime di «unanimità che è solo garanzia di inazione e impotenza», come ha tristemente ammesso il presidente del Parlamento europeo Borrell nel lasciare il suo incarico al neoeletto Pottering. Sul tavolo finora si sono formate e sono state avanzate tre ipotesi fondamentali. La prima è quella di mantenere il testo originale del Trattato a cui, caso mai, aggiungere elementi supplementari, ma senza nulla togliere all'impianto del Trattato in via di ratifica.

Andrew Duff, inglese, membro della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, nella sua «*Constitution plus*» scrive che il Trattato potrà sopravvivere solo apportando delle modifiche che tengano conto delle critiche espresse dall'opinione pubblica, la quale avverte il processo europeo penalizzante a causa, spesso, dell'eccessivo peso dei suoi vincoli e della sua burocrazia e troppo poco legato ad un profilo dell'identità e delle radici culturali e religiose. Nelle parti III e IV, le modifiche dovranno riguardare: la semplificazione delle procedure di revisione della parte III, con emendamenti miranti a modificare le politiche comuni e le loro disposizioni prevedendo una ratifica dei quattro quinti degli Stati membri; la ridefinizione della politica economica generale della UE adattata ai nuovi scenari della globalizzazione; il cambiamento degli obiettivi economici perseguiti dalla UE per includere e rafforzare le priorità della Strategia di Lisbona; l'istituzionalizzazione dell'Eurogruppo, con l'obiettivo di migliorare la *governance* economica della zona Euro e di accelerare le riforme strutturali degli Stati membri; da ultimo, ma non per importanza, la riforma della politica comune dell'energia per rispondere all'esigenza di sicurezza degli approvvigionamenti e per promuovere il ricorso a fonti di energia rinnovabili, senza tralasciare però la creazione di un nuovo capitolo sulla politica di allargamento che specifichi la procedura di adesione, definisca una nuova categoria di membri associati e rinforzi la politica estera. Richiamo, per la senatrice Gagliardi che è intervenuta prima, a proposito delle parole d'ordine per la pace e contro la guerra, le parole assai più significative di Angela Merkel nel suo discorso tenuto all'insediamento della Presidenza tedesca il 17 gennaio, e cioè che tutta l'Europa ha un fondamentale interesse al successo dello sviluppo dell'Afghanistan, così come l'Europa crede - e lo crede fortemente la Presidenza tedesca che solo la combinazione tra l'impegno militare e civile avrà successo, perché ogni altra iniziativa è destinata al fallimento. A noi più che le parole d'ordine colpiscono le parole chiave della semplificazione. Non ci stupisce che autorevoli *leader* come Nicolas Sarkozy in Francia e il ministro degli esteri olandese Verhagen si siano dichiarati disponibili alla negoziazione di un nuovo Trattato UE

la discussione diretta all'approvazione della risoluzione sul programma legislativo della Commissione europea è stata un'occasione molto importante per il nostro Parlamento e per il nostro Senato; debbo dirvi che, come tutti voi, ho potuto ascoltare, sia ieri in discussione generale,

abbia dato prova di vera consapevolezza dell'importanza dell'appuntamento che abbiamo davanti, appuntamento situato, come voi sapete, all'interno di una fase molto importante nella storia dell'Unione Europea. Noi oggi discutiamo tra il Consiglio europeo dell'8-9 marzo scorso e il prossimo appuntamento del 25 marzo, quando sarà celebrato a Berlino il cinquantesimo anniversario del Trattato di Roma.

l'occasione del Consiglio europeo, nelle riunioni dell'8 e del 9 marzo, quando il Cancelliere tedesco ha rilanciato la strategia di Lisbona e ha condotto a compimento una discussione strategica che ha portato a un accordo molto rilevante sulle questioni ambientali e climatiche, uno dei principali temi

Ho ascoltato con molto interesse - in modo particolare, nell'intervento del senatore Mantica - gli argomenti che sono stati portati

tempo: il processo costituzionale europeo. Nella prima Convenzione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonostante gli sforzi dell'allora presidente Roman Herzog, non fu adottata l'espressione «valori religiosi», senatore Mantica, ma si parlò di «patrimonio spirituale». Nella seconda Convenzione, presieduta da Giscard d'Estaing, fu adottata una prima formulazione che accoglieva un riferimento ai valori religiosi, ma

culturali, religiosi e umanistici dell'Europa. Questo complesso di richiami non è indifferente e merita di essere sottolineato, perché qualificava in qualche modo

porta le firme di Silvio Berlusconi, degli allora ministri Frattini e Buttiglione e, soprattutto, di Gianfranco Fini che rappresentava il nostro Governo presso la Convenzione presieduta da Giscard d'Estaing - si parlò di un'ispirazione riferita alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono poi sviluppati i valori universali di cui l'Europa stessa, nel suo complesso, si è fatta portatrice.

di Berlino il prossimo 25 marzo, in un testo che ormai mi sembra assolutamente consolidato, a meno che, come anche il nostro Presidente della Repubblica

1953 diceva, e vi leggo testualmente: «Ancora recentemente taluni hanno accusato noi sostenitori dell'Europa di stabilire nell'ombra una sorta di identità tra Europa e cristianesimo o, per meglio dire, tra Europa e cristianesimo tra Europa e cristianesimo cattolico. Prima ancora che infondata questa accusa è sciocca. Come concepire un'Europa senza tener conto del cristianesimo, ignorando il suo insegnamento fraterno, sociale e unitario? ricordare - concludeva De Gasperi - che il cristianesimo, essendo ai nostri occhi una cosa divina, appartiene e si indirizza a tutti gli uomini. Farne una cosa soltanto europea sarebbe limitarlo, sarebbe degradarlo». Credo allora che noi

con moderazione gli strumenti regolamentari, perché soltanto un uso moderato degli stessi può portare ai nostri lavori quel progresso e quel successo che meritano.

D'Andrea - che, dopo Berlino, potremo discutere in sede parlamentare? Abbiamo bisogno di dare oggi un'indicazione ai rappresentanti del Governo, perché Berlino sia uno snodo in cui essi possano farsi interpreti delle ragioni che emergeranno in quest'Aula.

Come si fa a dire che Berlino non sarà la tappa per fare il punto della ripresa del cammino europeo? Come si fa a non prevedere una sollecitazione al nostro Governo su questo punto specifico, che è, appunto, quello del riaffermare le radici giudaiche e cristiane dell'Europa? Saranno certo le elezioni europee - esse stesse - un *referendum* e potranno - quelle del 2009 tenere sveglie le coscienze, obbligando l'Europa a reagire. Riteniamo, signor Presidente, di essere impegnati nella ripresa del cammino europeo, riprendendo i riferimenti espliciti alle radici cristiane dell'Europa: un'Europa con una precisa identità culturale; un'Europa dei valori (che non nasce, da un relativismo senza princìpi, ma da valori che hanno plasmato l'identità europea nel corso dei secoli). Per queste ragioni, signor Presidente, mantengo l'ordine del giorno

Forse sono stato male interpretato: nessun impedimento all'allargamento. Quando poi il senatore Zanda parla di provocazione, ebbene, dico di sì. Questa è una provocazione nel senso di chiamare tutti a favore a favore di un pronunciamento. Riconoscere che una delle radici nel bosco dell'Europa è quella cristiana mi sembra un atto lapalissiano. Se poi, per qualche problema interno alla maggioranza, questo non può essere accettato perché c'è una sorta di scandalo il problema è vostro. Ma allora era provocatore anche il presidente della Repubblica Napolitano quando recentemente, il 20 novembre, ha parlato al Sommo Pontefice e ha detto: «Siamo convinti che molto possa fare per la causa della pace e della giustizia nel mondo l'Europa unita, parlando con una sola voce riconoscendosi in grandi valori condivisi, che riflettono il ruolo storico e la sempre viva lezione ideale del Cristianesimo». Questo non è Polledri, né Calderoli o Eufemi, ma è il presidente Napolitano.

più che geografici». Giuliano Amato riconosceva il valore identitario per l'Europa della religione cristiana e l'opportunità della sua inclusione. Ma sono tutti provocatori, o sono provocatori solamente perché non riuscite a dare una risposta semplice? Presidente, si sono inventati questo dibattito perché non avevano alcun argomento da portare in Aula. Ora questo dibattito sta prendendo una piega seria.

e alla propria coscienza. Non accettiamo però che tutte le volte che l'opposizione pone un argomento serio ci venga detto dagli eredi di Stalin che siamo dei provocatori. Questo deve essere ben chiaro! Voi non potete non sottoporvi ad un dialogo e ad un giudizio anche costituzionale e democratico. Pertanto, signor Presidente, ritiriamo gli ordini del giorno e convergiamo su una dichiarazione semplice

Le ragioni addotte contro l'opportunità di questo ordine del giorno infatti non ci convincono né da un punto di vista culturale né da un punto di vista politico.

poi non si possa ibridare e produrne degli altri. Affermare le radici giudaico-cristiane dell'Europa assieme alle radici greco-romane non significa negare l'importanza dell'Umanesimo, dell'Illuminismo e di quanto è seguito. Si tratta di un fatto, non di un'opinione, che chiunque e con qualunque fede politica dovrebbe avere la forza di riconoscere. Da un punto di vista politico non credo vi siano difficoltà o che si metta in pericolo la presidenza del cancelliere Angela Merkel nel momento in cui si afferma che vogliamo ripartire da questo dato. Significa solamente chiarire la consapevolezza dei motivi per i quali l'Europa fino ad ora è fallita. La cancelliera Merkel, intervenendo il 30 novembre 2005, si è così espressa: «Se rinunciassimo ai nostri valori, rinunceremmo a noi stessi». E l'11 marzo 2006 ha ribadito il concetto: «L'Europa si deve rifondare a partire da se stessa e mostrare in modo sempre più competitivo e globalizzato di sapere plasmare la politica secondo i propri valori». valori». Presidente, quello che noi dobbiamo affermare qui, oggi, è che le Costituzioni non cadono dal cielo; le Costituzioni rispondono a precise culture e solo se rispettano queste culture

facoltà per un minuto. Concedo i tempi che sono residuati rispetto alle dichiarazioni degli altri colleghi. intervengo solo per lasciare una traccia in un dibattito che rivela ancora una volta come questa maggioranza non voglia e non possa assolutamente

e si oppone a una discussione e a una votazione che noi invece ritenevamo normalissima. Nella scorsa legislatura, alla Camera, quando si discuteva - lei era presente, senatore Calderoli, a questi dibattiti politici nel Paese - di nuova Costituzione europea, nessuno scandalo veniva portato avanti quando si discuteva discuteva delle radici cristiane nella Convenzione, che vedeva presenti tra l'altro il senatore Dini, il presidente Fini e altri. Quindi, questa opposizione e questo pregiudizio rivelano quanto questa maggioranza sia prigioniera di un relativismo laicista che impedisce qualsiasi discussione su temi così ampi, fondamentali, nei quali tutto il Parlamento si dovrebbe riconoscere. Da qui la nostra posizione, che riconferma la posizione poc'anzi assunta dal senatore Mantica,

dal Vaticano sorgono messaggi sui valori che vengono interpretati come dissacranti verso il laicismo che, invece, pare imperare su questa maggioranza che vorrebbe che tale laicismo e relativismo incombesse su questo Paese. Da qui la nostra posizione,

riguardo all'ordine del giorno che richiama le radici cristiane dell'Europa, alcuni di noi - io per primo - si asterranno con questa motivazione.

la validità di una proposta che sul piano culturale è valida e per la quale i nostri rappresentanti in Europa, anche nella passata legislatura, hanno operato. Sentiamo le ragioni di una impossibilità, nell'auspicio che questo possa tradursi realmente in un risultato possibile, perché non possiamo assolutamente pensare che il Trattato costituzionale possa essere modificato. Quindi, la ragione della nostra astensione sta in questo: pur riconoscendo la validità dell'idea sul piano, non confessionale, ma meramente culturale, come riconoscimento di una radice culturale, riconosciamo altresì l'impossibilità che essa trovi una risposta concreta nelle procedure che attengono all'Unione Europea. Queste sono le ragioni per cui alcuni senatori si asterranno su questo ordine del giorno.

DISEGNO DI LEGGE Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere firmato a Roma il 27 novembre 2003, costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sull'aggiornamento della lista delle istituzioni culturali e scolastiche che godono di agevolazioni fiscali, con scambio di note integrativo, effettuato a Roma in data 28 luglio 2005 e 23 settembre 2005. Art. 2.

31 gennaio 2007 ho presentato un atto di sindacato ispettivo, l'interpellanza con procedura abbreviata